L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

della conformità della copertura del disegno di legge di bilancio alle regole stabilite in materia dalla vigente legislazione contabile. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente. «La Commissione programmazione economica, bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, premesso che: la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla disciplina contabile, che riguardano sia l'articolazione che i contenuti della manovra di finanza pubblica; per quanto riguarda l'articolazione della manovra, la novità più rilevante consiste nel fatto che sono stati accolti in un unico provvedimento (il disegno di legge di bilancio), composto da due sezioni, i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio) che, ai sensi della legislazione previgente, dovevano essere presentati alle Camere; in questo quadro, il disegno di legge di bilancio, sulla base di quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, non soggiace a una regola di copertura a una regola di equilibrio, per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare da esso risultante deve essere coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica; rilevato che, per quanto concerne i profili finanziari: la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare risultante dal disegno di legge di bilancio con gli obiettivi programmatici attraverso una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico; dalla tavola di raccordo emerge che, in corrispondenza di un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, pari a circa 39 miliardi nel 2017, 27 miliardi nel 2018 e 9 miliardi nel 2019, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni si attesta a circa 40 miliardi nel 2017, 20 miliardi nel 2018 e 3 miliardi nel 2019; tali valori del saldo netto appaiono coerenti sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2016, come modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra; esprime parere favorevole ritenendo che i valori del saldo netto da finanziate risultanti dal disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 siano coerenti con l'indebitamento netto programmatico risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2016, come modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra».

e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) è deferito alla Commissione bilancio in sede referente, con il parere di tutte le Commissioni permanenti, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

La Conferenza dei Capigruppo ha definito il calendario dei lavori. Le Commissioni permanenti dovranno rendere i propri rapporti alla Commissione bilancio entro le ore 20,30 di questa sera. Il disegno di legge di bilancio sarà discusso in Assemblea nella seduta unica di domani, a partire dalle ore 9,30. Gli emendamenti all'Assemblea dovranno essere presentati entro le ore 9,30 di domani. Come stabilito dal Regolamento, potranno essere presentati soltanto gli emendamenti respinti in Commissione. Qualora la Commissione bilancio non dovesse concludere l'esame del provvedimento, tutti gli emendamenti ivi presentati saranno considerati tecnicamente respinti. Poiché il Governo ha preannunciato di porre la questione di fiducia sulla Sezione I del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, la discussione in Assemblea sarà organizzata secondo le seguenti scansioni temporali. Dopo la relazione introduttiva e la votazione di eventuali questioni incidentali, è stato stabilito che in ogni caso le dichiarazioni di voto avranno inizio alle ore 12. Pertanto la chiama avrà luogo intorno alle ore 13,30. Dopo il voto di fiducia, si passerà alla votazione degli eventuali emendamenti e degli articoli della Sezione II del disegno di legge, nonché alla votazione finale con procedimento elettronico. Come da prassi, le dichiarazioni finali di voto si svolgeranno in un'unica fase, coincidente con le dichiarazioni di voto sulla fiducia.

dato un giudizio molto negativo nel merito di quella riforma costituzionale, ma anche delle politiche economiche e sociali del Governo (avremo poi modo e tempo di riflettere, non so se in quest'Aula o da altre parti, ancor di più sull'analisi e sul significato di questo voto). però che i cittadini si siano espressi (e con una certa chiarezza) anche nei confronti del metodo con cui il Governo ha proceduto sulla riforma costituzionale e che, ahimè, è stato una costante

dando vita, tra l'altro, a un inedito, perché ognuno di noi è andato a vedere se c'erano stati dei precedenti ed è un totale inedito quello di un Governo e di un Presidente del Consiglio che di fatto si è dimesso (sappiamo tutti che il Presidente della Repubblica gli ha chiesto di congelare le

per questo che siamo stati eletti, signor Presidente: per portare avanti le istanze e le proposte dei cittadini e rappresentare la sofferenza sociale

di metter mano a una manovra che, così come è, creerà non solo tanti problemi ai saldi e al bilancio dello Stato, ma ancora nuove criticità al nostro Paese.

Premesso che non esistono Governi tecnici, ma Esecutivi che, qualunque sia la loro composizione, ottengono la fiducia dal Parlamento e, quindi, la fiducia politica, a maggior ragione non possono esistere fiducie tecniche a un Governo politico che, nonostante le dimissioni annunciate dal Presidente del Consiglio, resta per ora, secondo la Costituzione, nella pienezza delle sue funzioni. C'è un altro argomento, signor Presidente, che vorrei sottoporle. Nel *referendum* di domenica, i cittadini italiani, quindi il popolo sovrano, hanno confermato una legittimazione piena al Senato della Repubblica. Io facevo parte del Comitato del Sì, ma devo prendere atto, inchinandomi alla volontà del popolo, che il Senato resta in questa legislatura e resterà nella prossima. Mi sembra perciò paradossale e scorretto che la legge di bilancio, la manovra di fine anno, che è l'atto più importante che il Governo fa e il Parlamento approva, sia liquidata dal Senato in quindici ore, senza possibilità di emendare,

Non si comprende questo comportamento, anche perché il nostro Gruppo, come molti Gruppi, si è limitato alla presentazione di pochissimi emendamenti, quelli ritenuti più importanti e che meritano davvero una discussione. Discussione, peraltro, già avviata alla Camera, con relazioni tecniche puntuali, per cui un esame approfondito Per tutte queste ragioni, come Gruppo, vorremmo procrastinare di due o tre giorni la discussione in Commissione per poi arrivare in Aula, quantomeno, con queste correzioni.

che domani la fiducia non venga chiesta da persone che hanno scritto la "schiforma" che è stata sonoramente bocciata dai cittadini: che abbiano almeno la dignità di fare un passo indietro.

per suffragio di popolo e a presidio di pubbliche libertà, il Senato della Repubblica rimane». il caso che la legge di bilancio, che è la legge più importante che quest'Assemblea licenzia durante l'anno, venisse esaminata con molta più attenzione di quanto non ci venga chiesto dal nostro Governo. Anche perché un dato fondamentale, che noi abbiamo ribadito in quest'Aula, è che c'è tutta una serie di poste che noi vorremmo tranquillamente verificare e, possibilmente, emendare. Peraltro, come ho già avuto modo di dire, siccome non mi appartengono le paternalistiche pietistiche del Presidente del Consiglio, il quale chiede sempre in nome dei figli, non avendone il sottoscritto e parlando, da parlamentare, nell'interesse del Paese, credo che l'interesse del Paese vada salvaguardato ed essendo il Senato nelle proprie funzioni, non possiamo licenziare una legge di bilancio che continua ad essere sempre rimandata con i costi al futuro. Avremmo necessità di salvaguardare l'interesse collettivo, di verificare e, ove possibile, di fare quei tagli necessari per evitare i rischi delle famose clausole di salvaguardia, che altro non sono che spese fatte da questo Governo nei due anni passati senza avere il patrimonio per poterle fare. quello di domenica è stato un voto che ci richiama alle nostre responsabilità e se dobbiamo assumere queste responsabilità, forse sarebbe il caso di iniziare a lavorare con un po' più di serietà e con meno pressapochismo, che questo Governo ha dimostrato fino ad oggi. Pertanto, mi associo alla linea dei colleghi nel chiedere che la legge di bilancio venga lasciata in Commissione in questi giorni e vada in Aula la settimana prossima. *(Applausi

coscienza di quello che si è detto per mille giorni, cioè il sogno di una "Renziland" dove tutto va velocemente, dove il Senato non esiste e dove lui non sarebbe più venuto qui a chiedere la fiducia. *(Applausi dal la prima cosa che disse il nostro attuale (e futuro ex) Presidente del Consiglio fu: io sarò l'ultimo Presidente del Consiglio che verrà in quest'Aula a chiedere la fiducia.

questo Governo e questo Presidente del Consiglio. Il bilancio dello Stato è talmente una cosa seria che è stato votato alla Camera, e considerato che

- esiste ancora il bicameralismo perfetto e di conseguenza, come abbiamo detto anche nella Conferenza dei Capigruppo, la stessa dignità che è stata data alla Camera dei deputati per poter trattare quel provvedimento deve essere data al Senato del Repubblica: quella dignità che merita questo provvedimento, quella dignità che merita quest'Assemblea e che meritano tutte le persone e tutti questi cittadini italiani che sono stati eletti da altri cittadini italiani per rappresentarli in quest'Aula, cosa che, ahimè, il Presidente del Consiglio, a cui manca la memoria, non ricorda mai. Signor Presidente, perché chiediamo

del preaccordo con i sindacati per quanto riguarda gli stipendi del pubblico impiego, la problematica dell'ILVA, le problematiche degli accordi tra lo Stato e le Regioni e la problematica degli accordi tra lo Stato e i Comuni,

è urgente, anche per far sì, come abbiamo consigliato al ministro Boschi, che l'opinione pubblica non pensi che quello che lui ha promesso durante la campagna elettorale, cioè i famosi soldi ai dipendenti pubblici, non sia la solita marchetta per portare a casa quattro voti in più. Portino a casa i risultati. Portate a casa quello che abbiamo promesso agli italiani.

che la prima promessa è stata: «Lascerò la politica». E ogni promessa è debito!

come membro della Commissione finanze. All'interno del testo ci sono diverse norme fiscali

la richiesta delle tasse a chi ha subito il terremoto, ma se pone la fiducia

rispettoso dei cittadini italiani, non può lasciare loro una legge di bilancio che li condizionerà il prossimo anno, senza avere nemmeno il tempo di leggerla, concedendo l'ennesima fiducia a questo Governo che nessuno vuole più. a tutti i parlamentari della maggioranza veramente di staccarsi da questo simbolo e da questa sudditanza a Renzi e pensare, per una volta, a cosa vogliono i cittadini italiani, ossia una legge di bilancio seria e non le solite

Grazie Comandante! Mi rifaccio a lei: mi ricordo che due anni fa, sempre in quest'Aula, per la legge di stabilità lei disse questa frase: «Adesso «Adesso approviamo la legge di stabilità e, dopo, la maggioranza la riscriverà». Credevo che in quell'occasione avessimo raggiunto il punto più basso, istituzionale, di questo Senato, oggi, in quest'Aula, iniziamo a scavare verso un punto ancora più basso, perché lei si prende la responsabilità di far approvare un disegno di legge bilancio che creerà negli enti locali un caos istituzionale senza precedenti nella storia dell'Italia: Comuni in dissesto, perché tutto quello che riguardava gli enti locali doveva essere discusso in quest'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Quindi, Comandante, l'altra volta fui io a dirle di tornare a bordo, questa volta gliel'hanno detto gli italiani: torni a bordo e si assuma una seria responsabilità

siccome il Senato c'è e rimane e lei è la seconda carica dello Stato, si assuma la responsabilità di far discutere questo disegno di legge di bilancio seriamente e di risolvere il caos istituzionale che altrimenti ne conseguirebbe. La responsabilità è tutta vostra, non di quelli che vengono dopo, come sempre; è vostra, che lasciate un caos infinito solo per l'economia delle marchette.

Signor Presidente, ella poco fa ha annunciato con la solita solennità l'apertura della sessione di bilancio;

Risparmio ai colleghi - anche perché molti l'hanno già evidenziato - il commento sul voto referendario. Saluto solamente quel voto con un «ben tornato, Senato»; ma è un ben tornato amaro, Presidente, perché è tornato a fare che? A sottostare ai *Diktat* di un Presidente del Consiglio, tra l'altro per ora abbastanza scombussolato scombussolato da un risultato che non si attendeva e che, invece, noi sapevamo essere nel sentimento dei cittadini italiani. però, siamo una forza responsabile, siamo convinti che l'esercizio provvisorio non sarebbe utile a questo Paese e vogliamo comunque salvaguardare la dignità di quest'Assemblea; non solo la dignità di questa Assemblea, ma anche gli interessi del Paese. Ricordo a me stesso prima ancora che ai colleghi che la legge di bilancio si forma in due letture e che, attraverso il dibattito in prima lettura, trova sbocco per alcuni provvedimenti importanti nella seconda lettura. I colleghi ne hanno ricordati alcuni: dall'ILVA di Taranto, ai provvedimenti per i Comuni, al rimpinguamento dei fondi utili per onorare il contratto (anche se chiaramente preelettorale)

avrebbe proposto a un Senato nel pieno della sua legittimità - non solo presente ma ormai anche futura - di dover votare una fiducia a un Governo che, invece, in questa legittimità non è più, avendo il Presidente del Consiglio detto chiaramente che le sue dimissioni sono politiche e irrevocabili, temporaneamente sospese solo per l'approvazione del disegno di legge di bilancio. Ma non del suo disegno di legge di bilancio. Costituzione, come recentemente novellato, impone al Parlamento di approvare la legge di bilancio anche se il Governo non dovesse essere più presente: quella è una discussione che potremmo portare utilmente avanti.

di previsioni non indispensabili, il che potrebbe aiutare - questa volta il Paese e non il Governo - ad affrontare meglio il giudizio dell'Unione europea. infatti sospeso l'interlocuzione con l'Unione europea; il ministro Padoan, dopo il risultato referendario, anche lui preso dal panico, non si è recato a Bruxelles. Da Bruxelles sono arrivati invece messaggi di apertura che ci invitano a risolvere la nostra crisi politica,

Noi vogliamo evitare che si parli di questo. Allora possiamo benissimo, in questi pochi giorni, eliminare gli appesantimenti della manovra che possono poi portare l'Europa alla richiesta perentoria di una manovra aggiuntiva e presentarci con un manovra pulita e stringata all'osso. Naturalmente il problema dell'IVA è quello che ci preme maggiormente in questo momento e siamo d'accordo che ne debba essere sospeso l'aumento dal 1° gennaio;

un termine infelice che si usa in queste ore, congelate per approvare la legge di bilancio, ma allora fu attivata una procedura ordinaria. A parte il fatto che in quel caso la caduta del Governo fu determinata non certo da un *referendum* così pesante come quello che si è svolto

è stata una scelta dettata dalla tracotanza di pensare che quel *referendum* sarebbe stato un ulteriore volano alle sue politiche. Quel *referendum* per fortuna invece è stato uno *stop* clamoroso

Riformulo una proposta già avanzata da altri colleghi, cioè quella di consentire alla Commissione bilancio di lavorare almeno questa settimana, festività compresa, come tante altre volte si è fatto, e di portare

parola greca *téchne*, che significa arte. La parola vuol dire perizia nel raggiungimento di un obiettivo. Nella dottrina costituzionale l'esempio di scelta tecnica trova

perché deve raggiungere l'obiettivo di non consentire che la durata della legislatura si protragga oltre il tempo e, quindi, la perizia nel raggiungimento dell'obiettivo lo sottrae all'obbligo costituzionale (ossia si scioglie il Parlamento quando è accertato il venir meno di una maggioranza). Nella dottrina costituzionale la perizia è quindi qualcosa che deriva dagli obblighi costituzionali. La fiducia tecnica è stata effettuata altre volte nel raggiungimento di un obiettivo costituzionale che non credo possa essere quello richiamato oggi dalla maggioranza e dal Governo, atteso che l'articolo 81 della Costituzione prevede che l'approvazione del bilancio sia un obbligo costituzionale che sottrae il Parlamento alla vita del Governo, così come viene sottratta alla vita del Governo la conversione dei decreti-legge. allora, che tutti noi sappiamo cosa sta avvenendo in quest'Assemblea. In quest'Assemblea sta avvenendo una compressione del diritto-dovere di ogni singolo senatore. Ogni singolo senatore ha infatti il dovere di fare le leggi,

In questo caso, qualora noi tutti accettassimo il calendario dei lavori così come voluto dal Governo e dalla maggioranza, verremmo meno a un nostro preciso obbligo, che è quello di "lavorare" il bilancio

dell'emiciclo sarebbe per me un grande successo - stiamo lavorando con un calendario che è soltanto, nel tempo, funzionale alla direzione del Partito Democratico di domani il bilancio prima della riunione della direzione, avrebbe tolto di mezzo uno dei motivi per cui la discussione potrebbe essere incentrata non sulle bramosie, sulle ambizioni, sulle presunzioni del Governo dimissionario, ma sul dovere che ha il Parlamento di procedere in un'attività legislativa che sia garanzia dello Stato, del popolo e del mandato ricevuto. Che sia ben chiaro: io sono contrario a questo calendario perché sono contro una ulteriore esposizione della nostra attività al ludibrio. Noi l'abbiamo esposta al ludibrio con il voto di fiducia sulla legge elettorale, con la votazione con la votazione di articoli premissivi che hanno stracciato e reso vana qualsiasi nostra attività per la modifica della Costituzione. *(Applausi dei Approvando questo calendario dei lavori, noi esponiamo ancora una volta al ludibrio il giudizio che poi, giustamente, in vena di antipolitica, il popolo dà alla nostra attività perché in questo momento non stiamo (dovrei

Signor Presidente, come ha spiegato bene il presidente Ferrara, è oggettivo il fatto che la nostra discussione e quindi la richiesta di porre la fiducia sul disegno di legge di bilancio è nient'altro che uno dei tanti atti legati alla faida interna al Partito Democratico. Quindi, ancora una volta, prendiamo in ostaggio le esigenze del nostro Paese perché ci possa essere un regolamento di conti all'interno del Partito Democratico.

perché alle 14,52 di oggi è avvenuto un fatto degno di nota: il Presidente neoeletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha comunicato, renzianamente via Twitter, che non intende più procedere all'acquisto del nuovo Air Force One, con un risparmio di 4 miliardi di dollari. Sarebbe bene, a questo punto, che noi inserissimo come emendamento nel disegno di legge di bilancio un saldo di fine stagione, cioè la vendita dell'Air Force Renzi e consentissimo 200 milioni di risparmi

avremmo un ottimo argomento per affrontare la campagna elettorale perché le nequizie che sono dietro all'acquisto di quell'aereo si sentiranno, sì, in campagna elettorale e ci consentiranno di scoprire perché, rinunciando alla dotazione dell'aeronautica militare, dobbiamo comprare aerei dagli arabi e da fondi come i fondi emiratini per coprire una lotta di potere che è un tutt'uno con le ragioni per le quali viene posta la fiducia domani mattina.

la fiducia, addirittura per fargli fare una legge che regolerà la politica economica dell'Italia. sarebbe forse opportuno lavorare come normalmente fa qualsiasi italiano in questa Nazione, quindi dalla mattina alla sera, anche di domenica, atteso che